Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 14, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Comunico che in data 2 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 30 novembre 2024, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Raffaele Fitto dalla carica di Ministro senza portafoglio. *F.to* Giorgia Meloni». Comunico, inoltre, che sempre in data 2 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, su mia proposta, con decreto in data 2 dicembre 2024, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. Tommaso Foti. *F.to* Giorgia Meloni». apre una nuova finestra"). Comunico che in data 29 novembre 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia*

l'immediata calendarizzazione di un intervento del Governo in Aula per riferire in ordine agli sviluppi della vicenda Stellantis che, come credo sia noto a tutti, ha conosciuto, nelle scorse ore, una situazione di forte tensione aziendale interna, con le dimissioni del capo aziendale e con una serie di procedure straordinarie che riguardano questa importante azienda, che ha una presenza industriale sull'intero territorio nazionale. Come i colleghi sanno, Stellantis è la struttura industriale che ha assorbito lo storico marchio della FIAT, che è stato il pilastro dell'industria italiana del Novecento. Novecento. Il tema dell'*automotive*, dal punto di vista produttivo, industriale e finanziario, va decisamente oltre il comparto in senso stretto, abbracciando una serie di casistiche dal punto di vista produttivo molto più ampie rispetto alla questione in sé, con un ruolo cruciale sul prodotto interno lordo, sull'occupazione, sull'innovazione del Paese e sulla sua capacità di essere presente nel quadro dei teatri mondiali. Peraltro, l'*automotive* oggi è il cuore di tre rivoluzioni che stiamo vivendo: la rivoluzione ambientale e climatica, che porta alla discussione sul motore elettrico,

subito e ai suoi massimi livelli, perché bisogna capire quali sono le misure, quali sono le politiche industriali, qual è la strategia e come si intende rispondere a questa situazione che rischia di avvitarsi con ripercussioni particolarmente negative all'interno del nostro Paese. La seconda è che l'azienda chiarisca immediatamente, perché ha una responsabilità sociale davanti al Paese, oltre che davanti ai mercati e ai propri azionisti e perché non può innescarsi una logica sulla base della quale i lavoratori vengono messi in cassa integrazione, ai *manager* si conferiscono le *stock option* e agli azionisti si assicurano i dividendi.

dobbiamo concentrarci sulla soluzione del problema. A urlare contro sono capaci tutti, ma poi i problemi rimangono sul tavolo e quindi abbiamo bisogno di creare condizioni favorevoli, in un contesto europeo molto complesso: leggiamo che cosa sta accadendo in Germania, con il marchio Volkswagen, che ha annunciato 15.000 esuberi; leggiamo di strategie industriali che riguardano Renault; leggiamo del rischio del blocco delle importazioni negli stati Uniti d'America sia per motivi legati alla sicurezza, sia per motivi legati al protezionismo nei confronti delle auto elettriche cinesi, con il pericolo che tutto questo si scarichi sul mercato interno europeo. Insomma, signora Presidente, credo, in conclusione, che ci siano sufficienti argomenti affinché il Governo riferisca prontamente anche perché il fatto che il primo Ministro venga a saperlo da una telefonata del presidente dell'azienda, senza informazioni preventive sul tema, ci pare un problema.

Camera, nonostante le proteste e le critiche avanzate da tutti i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione. Queste dimissioni evidenziano altresì la crisi gravissima attraversata dal settore *automotive* in Italia e in Europa. Non a caso, il 18 ottobre le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno proclamato unitariamente uno sciopero per denunciare questa crisi e l'assenza di risposte da parte della società e da parte del Governo. Presidente, il settore *automotive* è essenziale per il nostro sistema produttivo e l'economia del nostro Paese ed è attraversato da cambiamenti profondi. alla transizione ambientale: non si fa la decarbonizzazione, se non si interviene anche sulla mobilità, che è responsabile del 25 per cento delle emissioni di CO2. Pensiamo anche ai cambiamenti tecnologici: l'elettrificazione è molto avanti in alcuni Paesi, come pure la guida autonoma e sono in corso enormi investimenti da parte dei principali attori dell'*automotive* a livello mondiale. Questo settore in Italia, oggi, è segnato dal crollo della produzione di Stellantis di oltre il 30 per cento nel 2024. Siamo lontani anni luce dall'obiettivo di un milione di veicoli che era stato proclamato dal ministro Urso come credibile

tedesca e la crisi dell'industria automobilistica principale del continente, settore con cui le imprese, in particolare quelle del Nord Italia, sono fortemente interconnesse. Presidente, noi torniamo a ribadire in questa sede la richiesta che il presidente di Stellantis, John Elkann, che ha assunto un ruolo esecutivo dopo le dimissioni di Tavares, venga in questa

quando, a detta dei vertici della società, verrà individuato il nuovo amministratore delegato. Chiediamo però che anche il Governo venga di fronte al Parlamento e si assuma fino in fondo le proprie responsabilità. Nella legge di bilancio il Governo Meloni ha compiuto la scelta gravissima di tagliare dell'80 per cento il fondo *automotive* ereditato dal Governo Draghi, che scende da 5,8 a 1,2 miliardi: tali risorse erano destinate a sostenere la trasformazione e l'occupazione di un settore decisivo dell'industria italiana. Quel taglio è una decisione assurda, ancora più controproducente alla luce di quanto sta accadendo. si assuma le responsabilità, torni indietro su questa decisione insensata e si presenti al tavolo convocato il 17 dicembre con fatti concreti, a partire dal ripristino delle risorse e degli strumenti di politica industriale che sono indispensabili per affrontare questa crisi non a mani nude, ma con quello che chiedono le parti sociali del nostro Paese per aiutare un settore decisivo per la nostra economia.

un pugno in faccia ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese: la liquidazione di un *manager* che ha portato al fallimento l'azienda. Siamo di fronte al piano che aveva presentato due anni fa, che che è quello sostanzialmente di smantellare la produzione nel nostro Paese. Ora siamo di fronte a un buco nero e nessuno di noi sa come evolverà la situazione. Mi associo alla richiesta di

tutto l'indotto. Tutto il Paese viene coinvolto e quindi è necessario che questo Parlamento faccia una discussione di merito su qual è la politica industriale di questa grande

Non possiamo sottrarci, sperando che un giorno tutto si risolva, e chiedere solo gli ammortizzatori sociali. È necessario discutere di politica industriale, che non c'è nella proposta che si sta portando avanti. Insieme a questa ci sono anche altre crisi.

per quei lavoratori che per l'insieme del Paese. Mi associo e sostengo con forza la necessità che il Governo venga in Aula a discutere e che il presidente di Stellantis si renda disponibile a un confronto con il Parlamento italiano, perché deve rispondere soprattutto ai cittadini italiani. Signor Presidente, intervengo per aggiornare su quanto fatto non solo in Commissione, ma anche immediatamente dopo l'annuncio delle dimissioni del CEO Tavares del CEO Tavares rispetto alla questione Stellantis. Io e il presidente Gusmeroli abbiamo richiesto nuovamente al presidente Elkann di venire a riferire in Commissione sulla situazione attuale dell'azienda, anche alla luce del fatto che l'audizione di Tavares non ci aveva certo soddisfatto e credo che non avesse soddisfatto nessuna forza politica. Sin da subito tutti abbiamo manifestato l'intenzione di interloquire direttamente con la proprietà, per cercare di capire se esisteva un piano industriale e se quel piano industriale prevedeva la continuazione della produzione in Italia, visto che i dati già drammaticamente palesavano una situazione assolutamente differente da quella che Tavares aveva

Tavares allora disse al ministro Urso che, a fronte di queste due operazioni, avrebbe garantito la permanenza della produzione dei veicoli in Italia, che avrebbe raggiunto e mantenuto il milione di unità. nel 2024 è assolutamente impossibile, perché probabilmente non si raggiungeranno nemmeno i 400.000 veicoli prodotti, e manifesta l'incapacità dell'azienda di leggere la situazione attuale, travolta da una serie di operazioni che Tavares ha fatto nel breve per capitalizzare velocemente anche un interesse squisitamente personale. Ricordo a tutti che i dati disponibili raccontano di un CEO di Toyota che riceve un compenso di 10 milioni di euro, di quello di Volkswagen che ne riceve 9 e di un Tavares che l'anno scorso, senza la buona uscita di 100 milioni,

che ha visto nascere Stellantis, noi chiedevamo il *golden power* da parte del Governo, ma anche la partecipazione societaria, cosa che la Francia ha fatto e che oggi la porta ad avere

oggi i brevetti depositati in Francia sono almeno cinque volte superiori a quelli presentati in Italia. Ciò a dimostrazione di una capacità da parte della Francia di leggere la situazione già allora, cosa che non è accaduta qui, mentre i toni trionfalistici dei Governi di allora avevano visto la nascita di Stellantis come la panacea di tutti i mali. Noi già allora segnalammo il grande problema e già allora facemmo presente che, senza un preciso e puntuale da parte del Governo italiano, sarebbe stato difficile mantenerla, anche alla luce dell'ideologia assurda che, per per non rimanere sulle fonti fossili, porta tra le braccia di chi oggi ha sviluppato una tecnologia molto prima di noi, e cioè la Cina, facendo di fatto passare da una dipendenza ad un'altra. Oggi l'indipendenza dell'azienda automobilistica italiana è pari a zero, quindi il Governo fa bene ad aspettare il piano industriale di Stellantis e a capire quali sono le iniziative che intende mettere in campo. Ricordo a tutti che durante l'audizione, su richiesta mia e del senatore Calenda, chiedemmo di vedere il piano industriale

che Elkann venga in Commissione, sia audito dalle forze politiche e dimostri l'attaccamento che qualche forza politica crede che lui abbia nei confronti dell'Italia, ma che mai ha dimostrato, per farci vedere un piano industriale serio, in base un Governo serio faccia una seria politica non solo industriale, ma anche di tutela dei lavoratori.

Ci sono gruppi tedeschi e svedesi che hanno annunciato la chiusura di stabilimenti, mettendo per strada decine di migliaia di dipendenti in Europa. Su questo scenario, che ha responsabilità politiche ben chiare e che non dobbiamo dimenticare, si innesta poi la vicenda Stellantis, cui amministratore, che abbiamo audito qualche settimana fa, ha tenuto un atteggiamento di prosopopea e di arroganza nei confronti di tutto il popolo italiano che non ha precedenti.

stato risposto, con un atteggiamento di un'intolleranza insopportabile. Aggiungo, come ricordava il presidente De Carlo, che il nostro presidente Gusmeroli ha chiesto più volte l'audizione del presidente Elkann, che adesso diventa indispensabile indispensabile per capire qual è il piano industriale di questo gruppo, che ha tratto vantaggi dalla storia automobilistica italiana e non permetteremo che ne rappresenti la fine.

molto contenti di poter fare domande. Aggiungo però un elemento, Presidente, su cui certamente non saremo d'accordo, perché c'è un fantasma che aleggia su questa discussione e che ogni tanto si palesa sullo scalone di via Veneto al Ministero delle imprese e del depredato totalmente il fondo *automotive* di 8,7 miliardi (è un dato diverso da quello che indicava il senatore Misiani) con il decreto n. 17 del 2022, che ha consentito una politica industriale di taglio totale di ogni tipo di incentivo alle imprese italiane. È il fantasma del ministro Urso *(Applausi)*, che deve venire in quest'Aula a dirci sia qual è il suo piano industriale per l'*automotive*, sia - di grazia - anche qual è il piano industriale per il Paese, perché non ce n'è traccia. ancora una volta le sorti di un gruppo industriale fondamentale nella storia italiana si incrociano con preoccupazioni occupazionali e in prospettive di carattere più generale. Anche il Gruppo Forza Italia ha giudicato sprezzanti e inaccettabili alcuni atteggiamenti nei confronti del Parlamento e delle istituzioni da parte del gruppo Stellantis, ma al di là delle discussioni che in queste ore richiamano l'attenzione, ho condiviso le parole del segretario della CISL Sbarra, che sta dimostrando grande saggezza e concretezza, in linea con le tradizioni del sindacato che guida, nel dire che questo amministratore non ci mancherà. Non abbiamo visto risultati fantasmagorici e siamo come tutti esterrefatti di fronte ai compensi finali di cui si favoleggia, che saranno pure frutto di accordi contrattuali, tuttavia bisogna anche valutare i risultati. Certi *manager* vengono superpremiati quando i risultati sono importanti e forse alcune stagioni lo sono state. Avrà meritato anche risultati brillanti,

questo esborso. L'occasione per il nostro Gruppo in questa discussione, oltre a chiedere tutti i confronti in Parlamento con il Governo e con lo stesso gruppo Stellantis, è però quella di fare nostro l'impegno che il Partito Popolare Europeo ha animato: bisogna rivedere le date europee di passaggio all'auto elettrica; bisogna smetterla con la demagogia iper-ambientalista. Noi abbiamo un'agenda europea che, soprattutto per le pressioni di Timmermans e dei Gruppi socialisti, ha scandito traguardi impossibili: l'auto elettrica nel 2035, la casa *green* a spese degli italiani (invece il superbonus, casomai, premiava i furbi). furbi). C'è tutta un'agenda europea da ridefinire. Siamo lieti che la vicenda inevitabilmente complessa della Commissione europea abbia avuto epilogo. La Commissione europea ha inevitabilmente una formazione eterogenea, perché si tratta di 27 Paesi con Governi diversi: tutti devono stare nella Commissione e non possiamo aspettarci che tutti i Governi europei siano moderati o progressisti, liberali o socialisti. Quindi, la costruzione della Commissione europea è stata inevitabilmente complicata. L'Italia ha peraltro conseguito un ruolo autorevole che prima non aveva, con un Vice Presidente con deleghe esecutive. Ora, fermo restando l'obiettivo di un mondo meno inquinato e con industrie, automobili e palazzi meno inquinanti,

emesso nel mondo. Pertanto, non dobbiamo avere un complesso di colpa. Ci sono piattaforme continentali che inquinano in maniera mostruosa. In questo momento sulla crisi dell'industria automobilistica, al di là dei giudizi, che pure daremo,

da socialisti alla Timmermans o addirittura dalle Greta Thunberg, ma dalla realtà. Per avere sviluppo industriale dobbiamo correggere l'agenda europea e quelli che hanno causato questo disastro non possono fare la lezione agli altri.

recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali***

Signor Presidente, devo purtroppo riferire che non ci sono stati i tempi tecnici per poter concludere l'*iter* del provvedimento in Commissione. Pertanto, non è stato votato il mandato al relatore. finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 1310, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione,

in questo caso - come in tanti altri - del tutto privo dei prescritti requisiti di necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Su 4 leggi approvate dal Parlamento, 3 hanno matrice governativa e di esse circa il 40 per cento è costituito da conversione in legge di decreti-legge. L'azione di questo Governo - è successo anche altre volte in passato, ma qui davvero raggiungendo, purtroppo, le vette più alte - si contraddistingue per una serie di forzature sempre più evidenti al sistema legislativo, per l'esautoramento di fatto del Parlamento e per la vera e propria torsione dei principi costituzionali. In questo caso specifico, con questo decreto-legge, si prosegue sulla via di un pericolosissimo conflitto istituzionale con la magistratura, il tutto per alimentare una perenne campagna elettorale, nella fattispecie - come spesso succede - sulle spalle dei migranti. Peraltro, quando la Presidente del Consiglio - come ha fatto anche recentemente - afferma che sui migranti decide il Governo, io vorrei sommessamente ricordare che sopra a tutto non c'è il Governo, ma c'è la legge. Ed ancor sopra la legge c'è la Costituzione *(Applausi)* e ci sono i principi internazionali di rango costituzionale. Il Governo, anche questo Governo deve attenersi a questi principi. Invece, il testo del decreto in molti dei suoi punti si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale,

la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni di italiani sono partiti per l'estero nel periodo tra l'Unità d'Italia e i primi decenni i primi decenni del secolo scorso. Quasi sei milioni sono quelli che oggi vivono stabilmente all'estero. Il decreto contiene molteplici modifiche in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori, protezione internazionale speciale, diritto di asilo, procedure di espulsione e respingimento, con una notevole complessità degli istituti coinvolti. Ciò avrebbe dovuto evidentemente essere oggetto di una proposta di legge ordinaria, non foss'altro per valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali. Risultano, invece, particolarmente preoccupanti, anche sotto il profilo e il versante costituzionale, le disposizioni in materia di limitazione, divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale. Qui è chiarissimo il riferimento a una autentica ossessione del Governo, e cioè le imbarcazioni delle ONG che nel Mediterraneo operano - ricordiamolo sempre - solo al fine di salvare vite umane e che invece vengono nuovamente penalizzate nel loro diritto *(Applausi)*, introducendo una riduzione significativa, molto significativa, dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave da sessanta a dieci giorni. Questa disposizione, dal nostro punto di vista, è in palese contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde a un obbligo etico e morale di civiltà millenaria, oltre che a un obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio. Ancora, è molto grave quanto viene previsto ai fini, della identificazione dei migranti, dell'accesso ai loro dispositivi elettronici e digitali. Tale ispezione verrà disposta dal questore senza autorizzazione della magistratura e consisterà nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedente la protezione internazionale. Tutto questo - a nostro avviso - è in palese violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, principio sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15; il quale articolo aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; ma anche in realtà, in violazione del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione medesima, che recita che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. È recente la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, che afferma che lo scambio di messaggi elettronici rappresenti di per sé una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione. È illegittimo anche - dal nostro punto di vista - l'articolo 12-*bis* del decreto-legge, che definisce per legge l'Egitto e il Bangladesh Paesi di origine sicura, ignorando che lo scorso 4 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta proprio sulla definizione del Paese sicuro e ha specificato che un Paese è considerato sicuro se, sulla base dello *status* giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e uniformemente persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano e degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale. Io ve l'ho detto più volte in quest'Aula ve lo ripeto altre volte: la sola memoria di quanto successe a Giulio Regeni dovrebbe essere per tutti quanti noi una ferita ancora aperta, da non archiviare così miseramente. *(Applausi)*. Presentano inoltre profili di incostituzionalità anche gli articoli 13 e 14 sulle domande di protezione internazionale. L'articolo 14 prevede addirittura che, in caso di mancata presentazione del richiedente, la commissione possa non solo sospendere la domanda, ma deciderne il rigetto; ancora, appare del tutto criticabile la decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contratti, che sembra rivelare - in questo caso credo abbastanza palesemente - come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania è meglio vada nascosta. È molto grave, in questo senso, l'attacco portato alle sezioni specializzate dei tribunali, con l'obiettivo di mettere da parte i giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. Queste norme sono un tentativo - secondo noi palese di demolizione di alcune garanzie procedurali a tutela dei migranti; in particolare un attacco gravissimo agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana; attacco che peraltro mette evidentemente in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Come si vede - come ha dimostrato anche il caso Albania - le politiche che il Governo ha perseguito in tutti questi mesi - molti decreti-legge sono stati varati in questi mesi, come sappiamo sembrano rispondere più a esigenze di insopportabile propaganda sulle spalle dei migranti, che non a ragioni effettivamente di necessità. In conclusione, il decreto-legge in che questo Governo porta avanti, in particolare sulle politiche che riguardano la migrazione, delle scelte che nulla hanno a che vedere con la regolamentazione dell'immigrazione e che, non foss'altro che per questa ragione, ci vedono molto contrari. È un decreto-legge - a nostro avviso - incostituzionale e per questo chiediamo al Parlamento di votare a favore delle questioni pregiudiziali presentate.

di non procedere all'esame del decreto-legge in esame, cosiddetto decreto flussi. Io non entrerò in tecnicismi che sono incomprensibili al di fuori di quest'Aula,

assolutamente nulla. Solo nel mese di novembre sono stati 8.000 gli sbarchi, 64.000 gli sbarchi nell'anno precedente, per non parlare del *record* negativo assoluto toccato durante il 2023. C'è un filo che lega tutti questi interventi - anche il decreto presente - che noi chiediamo - ripeto - di non esaminare: è la convinzione che, mostrando un volto truce

ottenuto, invece, con l'ossessiva prosecuzione su questa strada? Una cattedrale nel deserto costruita in Albania, dove i nostri agenti di Polizia sono costretti, nella noia, a fare la guardia Questa è l'umiliazione a cui avete sottoposto i nostri agenti delle Forze dell'ordine, di cui pure tutti i giorni vi riempite la bocca, ma ai quali vi guardate bene dal dare vero sollievo e solidarietà attraverso misure concrete, come maggiori assunzioni o aumenti degli stipendi. I nostri agenti di Polizia sono soli nella noia e hanno fatto, a quanto pare, un atto di estrema umanità, accogliendo i cani all'interno di quel carcere che rimane vuoto. Perlomeno la la propaganda i partiti di maggioranza dovrebbero pagarsela con i soldi propri, e invece se la pagano con i soldi dei contribuenti. *(Applausi).* Guardate, non c'è niente di male nella propaganda, siamo abituati alla vostra propaganda. Ma almeno abbiate la dignità di pagarvela con i vostri soldi e non con i soldi degli italiani e delle italiane, che già se la passano male. Cosa prevede questo decreto? Ulteriore compressione dei diritti dei migranti con la violazione della *privacy*, con la compressione ulteriore, che già era stata fatta, del diritto anche internazionale e umanitario dei salvataggi in mare, quindi limitando e rendendo ancora più difficoltose e complesse le operazioni di salvataggio; volto truce sperando nella deterrenza: una strategia crudele, inumana e fallimentare. Cos'altro prevede Vedete, colleghi, questa maggioranza ci ha abituati al fatto che quel volto truce non lo mostra soltanto all'esterno, ma lo mostra anche all'interno, verso le stesse istituzioni. Vogliamo dire perché non ci sono stati i tempi tecnici per l'esame di questo decreto-legge, presidente Balboni? Si viene in Aula e si dice che non ci sono stati i tempi tecnici e le persone fuori da qui pensano da chissà cosa dipende, se da qualche casualità o da una congiunzione astrale. Ma il fatto che non ci siano stati i tempi tecnici perché il Governo non consente i tempi tecnici *(Applausi)*. Il Governo ha umiliato per l'ennesima volta il Parlamento e la Commissione affari costituzionali, addirittura mettendo sotto

per magia adesso diventa un emendamento che infiliamo nel decreto flussi alla Camera, quindi con conflitto di competenza e con umiliazione di questa istituzione che anche i colleghi di maggioranza dovrebbero rappresentare. ma non funzionerà, perché le istituzioni hanno gli anticorpi adatti per contrastare i vostri attacchi squadristi. Proprio oggi avete ricevuto l'ennesimo schiaffo sull'autonomia differenziata dalla Corte costituzionale, che ne ha smontato ogni pezzo, dimostrando non solo che le che le istituzioni che voi state cercando di indebolire ed attaccare hanno gli anticorpi adeguati a contrastare i vostri attacchi, ma anche che è l'Italia che ha gli anticorpi adeguati a contrastare i vostri attacchi squadristi che mettono in discussione le istituzioni, la Costituzione e le regole della convivenza civile in questo Paese.

Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, è stato ricordato

Siamo di fronte ad un uso smodato e ingiustificato della decretazione d'urgenza. Nel caso di specie, il decreto-legge n. 145, che è stato pubblicato l'11 ottobre e che deve essere convertito entro il 10 dicembre, rappresenta forse - anzi direi certamente - un provvedimento *record*. *record*. Francamente non ricordo un altro provvedimento così pieno di disastri e fallimenti sul piano della procedura Se dovessi fare l'elenco di tutti i principi che vengono fatti a pezzi da questo provvedimento, esso occuperebbe tutto il tempo che ho a disposizione per illustrare la questione pregiudiziale. Mi limiterò soltanto ad alcuni esempi. Il provvedimento è fallimentare sul piano dei contenuti perché viola in più parti articoli della nostra Costituzione, tra i quali - come è stato già Ostacola qualsiasi intervento serio di soddisfacimento delle esigenze che le imprese italiane hanno più volte manifestato, per quanto riguarda la carenza di manodopera in alcuni ambiti della nostra economia, altresì i ricongiungimenti familiari. Fa di tutto per creare problemi ai percorsi di integrazione di chi già si trova sul nostro territorio, magari da tanto tempo. Contiene quella norma particolarmente odiosa e disumana, oltre che in contrasto con la Costituzione, che riguarda la possibilità, senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di accedere ai dispositivi elettronici dei migranti che arrivano nel nostro Paese e fanno richiesta di protezione internazionale. Questi sono soltanto alcuni dei punti che, sul piano del merito, prestano il fianco a molte critiche e fanno anche capire, dato che siamo di fronte all'ottavo decreto-legge che il Governo fa su questa materia - è quella che è stata chiamata da alcuni colleghi una ossessione; termine che trovo adatto, perché siamo evidentemente di fronte a una fissazione, alla mania di produrre norme su un argomento *(Applausi)* a gettare in pasto all'opinione pubblica *slogan* ai quali non segue niente, con l'intento non di risolvere un problema, ma di strumentalizzarlo a fini di consenso

è un provvedimento matrioska: così chiamano gli studiosi i decreti-legge nei quali surrettiziamente vengono fatte confluire norme di decreti-legge emanati successivamente. Stavolta la vittima di questa confluenza surrettizia e ingannevole è stato il Senato della Repubblica, al quale è stato impedito di esaminare il provvedimento, e non soltanto perché esso è arrivato nella nostra Commissione a sette giorni

dando un'ulteriore prova di disprezzo verso l'istituzione parlamentare che, a questa forma di disprezzo, dovrebbe opporre una reazione unitaria. Non mi stanco mai di dire tutte le volte che intervengo su questo argomento che lo schiacciamento delle prerogative del Parlamento ad opera del Governo riguarda tanto l'opposizione quanto la maggioranza. Anche Anche i parlamentari di maggioranza dovrebbero conservare la volontà e il desiderio di indignazione nei confronti di una tecnica di produzione normativa così palesemente sgangherata e offensiva delle prerogative parlamentari. Però i nostri appelli, da questo punto di vista, continuano a cadere nel vuoto. Siamo di fronte a una maggioranza che, qualsiasi cosa faccia il Governo, anche la più offensiva del Parlamento, si mostra supina e accondiscendente e lascia passare tutto, dimenticando le cose che ha detto sulla centralità del Parlamento quando era opposizione. Vorrei infine dire altre tre cose per cui il provvedimento non dovrebbe essere oggetto di ulteriore esame da parte di questa Assemblea. La prima è una riflessione

che tutti i contribuenti italiani stanno pagando a caro prezzo. Credo che alla fine certificheremo che c'è stato uno spreco di centinaia di milioni di euro. è chiaro perché volete mettere il bavaglio alla Corte dei conti: avessi anch'io combinato le cose che state combinando voi, il desiderio di mettere il bavaglio alla Corte dei conti certamente farebbe parte

ciò che è stato fatto, da parte del Governo e della maggioranza, in termini di contrapposizione con il diritto europeo e con la giurisprudenza europea. Quando avete dovuto prendere atto che le norme emanate dovevano essere disapplicate, perché in evidente contrasto con il diritto comunitario e con la giurisprudenza comunitaria, avete completamente perso la tramontana, dando vita all'emanazione di un altro provvedimento, facendolo sparire dal Senato e facendolo riapparire alla Camera sotto forma di emendamento (come in un gioco di prestigio), perché ci fosse poca possibilità di esaminarlo e di approfondirlo. c'è stata tutta la pantomima della guerra lanciata contro i giudici delle sezioni dei tribunali specializzate sull'immigrazione. Ci sono dei giudici che fanno delle sentenze sgradite al Governo? Come in ogni brava democratura che si rispetti, non si pensa a cambiare il provvedimento, ma si cerca di cambiare il giudice. sezioni specializzate, dove ci sono dei magistrati che hanno approfondito l'argomento e che sono molto preparati sul tema, si toglie loro la competenza su questa materia per affidarla alle corti di appello, che in gran parte, tramite i loro presidenti, vi hanno detto che questa decisione è irrazionale, in quanto essi non hanno né le risorse, né la specializzazione, né la possibilità di affrontare questi contenziosi in maniera ordinata e razionale. Ma in fondo a voi di affrontare in maniera ordinata e razionale le cose non importa niente. Si continua a procedere a colpi di forza. I numeri che avete in Parlamento vi consentono qualsiasi tipo di esagerazione e di eccesso. Credo che l'uso anomalo e smodato dei decreti-legge resterà nella storia come una cosa davvero deprecabile e come una pagina nera della storia parlamentare del nostro Paese. Noi continuiamo a farvelo

Prima di passare alla discussione sulla questione pregiudiziale, voglio ricordare che, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, domani saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità (conflitti di attribuzione, casi Giovanardi e Sudano). Visto che ho fatto questo annuncio, ne faccio uno di altra natura. Oggi è il compleanno prima di tutto del presidente Casini. Facciamogli un applauso.

e ultimo, ma non ultimo, del mio amico Roberto Menia, e non che gli altri non siano amici.

troppo buono. Grazie. Torniamo a noi. Io e il mio Gruppo voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità, perché riteniamo che questo decreto-legge faccia carne da cannone della nostra Carta costituzionale, a partire da uno degli articoli fondamentali, l'articolo 70, che così recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

che ha letto dai giornali o che ha deciso di studiare durante il fine settimana. Questo decreto è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati il 27 novembre, che - se non vado errato - era mercoledì o giovedì scorso; oggi è martedì, la seduta è appena cominciata e noi siamo già in Aula con un provvedimento che questo Senato non ha potuto conoscere, non ha potuto discutere, non ha potuto modificare. È un provvedimento che il Senato si appresta a ratificare subendo una umiliazione che credo vada lasciata negli atti del Parlamento, e compiendo un atto di sottomissione al Governo, che legifera sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, che il Parlamento converta in legge, secondo il normale procedimento legislativo, quelle che sono decisioni prese su due piedi, rapidamente, in un Consiglio dei ministri. Tutto questo avviene con un decreto-legge molto corposo di svariate decine di articoli - credo siano ventuno o ventidue articoli - che incidono pesantemente sullo stato di libertà di persone che sono portatrici di diritti riconosciuti

trasceso, sia andato al di là delle sue potestà costituzionali. E credo si stia configurando in capo a ciascuno di noi, colleghi e colleghe, una violazione delle nostre prerogative di legislatori. *(Applausi)*. Si dice che si debba conoscere per poter deliberare: tutto questo non accade. Penso che il Presidente del Senato, che tra le altre cose è responsabile di tutelare l'onorabilità e le funzioni di quest'Assemblea, debba farsene carico. In secondo luogo, c'è l'articolo 77 della Costituzione che ho appena citato, che è quello che delega, in circostanze straordinarie di necessità e urgenza

forse uno degli elementi - la mobilità, il villaggio globale nel quale il nostro pianeta si è trasformato - caratteristici del nostro tempo. Noi ci troviamo davanti a una drammatica crisi demografica. Sappiamo bene che, nel giro di quindici anni, abbiamo perso 200.000 nascite e si si prevede che nel 2024 in Italia saranno nati meno di 300.000 bambini. Quello che ci si aspetterebbe da una classe dirigente responsabile è di mettersi a un tavolino Ferro: se il Ministro Schillaci ha appena fatto un accordo per portare in Italia 10.000 infermieri dall'India, perché questo è ai margini del G20 - il ministro Schillaci è andato dal Ministro della sanità indiano e ha chiesto non uno, non due, non 10, ma 10.000 infermieri dall'India - vorrà dire che siamo arrivati a un punto nel quale noi, come italiani, non riusciamo a coprire delle posizioni fondamentali per il funzionamento del Paese. Se così non fosse, non andremmo a chiedere all'India di mandarci 10.000 infermieri. ci aspetteremmo dal Governo una sessione straordinaria del Parlamento per discutere come si utilizza questa straordinaria opportunità che è la mobilità da da Paesi dai quali fuggono tantissime persone verso Paesi dove la manodopera è richiesta come il pane; basta andare a chiederlo ai nostri imprenditori. Invece voi ci fate un decreto-legge come fosse un terremoto, un'alluvione o una cosa imprevedibile. È evidente che questo decreto-legge non è stato emanato in ossequio e in applicazione dell'articolo 77 della Costituzione. Poi c'è una serie di violazioni di violazioni "puntuative" che, anche lì, strame di alcuni principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Faccio un esempio: l'articolo 25 della Costituzione dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Che cosa fa un Governo che decide improvvisamente che un certo giudice (leggi: le sezioni specializzate dei tribunali in materia migratoria) non gli piace, che sicuramente è il giudice naturale precostituito per legge? Fa una legge per cambiare quel giudice che non è più naturale. Naturale non vuol dire che sta in natura: vuol dire che è il giudice previsto naturalmente dall'ordinamento. Il giudice che voi scegliete oggi, quello delle Corti d'appello, è artificiale, non è naturale, perché è una decisione presa in modo reattivo rispetto alla giurisprudenza del giudice naturale. Dove lo mettiamo l'articolo 25? Chiedo al Governo. Poi, vogliamo parlare dell'articolo 31? Qui ci riempiamo la bocca della famiglia, dell'infanzia, eccetera.

Vogliamo parlare dell'articolo 15, quello che dice che la libertà e la segretezza delle comunicazioni, di qualsiasi genere, sono preservate dalla Repubblica? E che per violare quel principio ci vuole un provvedimento dell'autorità giudiziaria? Anche a questo articolo della Costituzione diciamo arrivederci, o forse addio, perché, sempre tramite decreto-legge che il Parlamento nemmeno può esaminare (perché viene letto, modificato e approvato da una Camera sola e ratificato dall'altra), si decide che, grazie al questore, si può guardare guardare nei telefonini delle persone. Mi fermo qui perché il tempo è finito, ma la lista di articoli che avete violato con questo decreto non finisce certamente

prima fra tutte quella un po' più cliccata, se vogliamo rimanere nell'argomento del decreto flussi, della mancata urgenza.

questo Governo è il primo che ha aumentato in maniera significativa i flussi regolari. Chi parla oggi di agevolarli aveva previsto numeri di flussi regolari molto inferiori a quelli fatti da questo Governo

regolari, si è accorto di qualcosa di cui nessuno si era mai accorto, o che forse nessuno si era mai preso la briga di controllare. Sui flussi regolari esisteva un vero e proprio sistema di frodi, con immigrati che pagavano delle somme per lavori che non venivano mai richiesti ed eseguiti. Era un vero e proprio traffico di permessi di soggiorno. Quel giorno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alla Procura nazionale antimafia e oggi quel procedimento, quel procedimento, che è andato avanti, vede diversi indagati. Questa è una delle ragioni essenziali

quella legale e regolare, il primo passaggio è mettere fine all'illegalità che c'è stata sino a oggi in questo Paese e che la sinistra non ha mai voluto guardare. *(Applausi)*. Questa è la verità e questo è uno dei principali motivi dell'urgenza di questo provvedimento.

il tema dei flussi e il tema dei Paesi sicuri, particolarmente dibattuto, rientrino perfettamente nelle prerogative del nostro Stato. Tra l'altro, ne sono stati tolti tre dalla lista dei Paesi sicuri.

dobbiamo essere in grado di scegliere chi entra in Germania. Macron dice che la nuova legge sull'immigrazione è lo scudo che mancava e che bisogna battersi contro i flussi illegali. Starmer

sono fuori dall'Europa, sono fuori dal mondo: non le sostiene più nessuno queste politiche migratorie senza controlli.

continuare a parlare della redistribuzione dei migranti. È l'unica grande soluzione che siete in grado di proporre, che è come proporre a un regista di come proporre a un regista di produrre un film muto e in bianco e nero nel 2024, quando esiste lo *streaming*. Non parla più nessuno in Europa di redistribuzione. Tutti parlano di difesa dei confini e ci sarà una ragione se gli altri Paesi guardano a questo modello con attenzione e iniziano a e iniziano a implementare le politiche contro l'immigrazione. *(Applausi).* Per carità, noi accettiamo i controlli giurisdizionali. Crediamo che sia legittimo lamentarsene. Mi fa un po' sorridere che la sinistra abbia sempre bisogno dell'aiuto da fuori. Una volta c'era la trasmissione Chi vuole esser milionario, dove si chiedeva l'aiuto da casa. Chi vuole essere rivoluzionario, invece, chiede l'aiuto al tribunale, sperando che qualcuno

Ritengo che sia la dimostrazione che questo Governo ha individuato nel contrasto all'immigrazione clandestina una priorità e, nella promozione dell'immigrazione irregolare, un'altra priorità. decreto al nostro esame non ci sono soltanto restrizioni, ma ci sono importanti normative per cercare di contrastare il caporalato, per andare incontro ai lavoratori regolari e per mettere delle quote per le donne. Ci sono tanti pezzi di normativa che riguardano proprio chi viene

Purtroppo, vi diamo quella che è una brutta notizia per voi, ma che è una buona notizia per l'Italia: i dati ci dicono che nel 2024 gli sbarchi sono calati del 65

intervenga sul tema dell'immigrazione. *(Applausi)*. Ve lo dico perché capisco la malinconia della sinistra per i bei tempi nei quali si parlava di redistribuzione, come ho detto prima. Capisco che la sinistra forse rimpianga la mangiatoia dell'accoglienza che c'era quando c'era l'immigrazione diffusa, quando le cooperative mangiavano e non garantivano niente a questi immigrati e oggi ci si aggrappi a 8.000 euro, perché questo è il costo reale di utilizzo della nave che porta e porterà i migranti in Albania. Fatevene una ragione: il centro il centro in Albania funzionerà e anche in questo caso le vostre previsioni verranno smentite dai fatti, come sono state smentite tutte quelle attuali. Capisco anche lo sconforto della sinistra per aver infranto il suo sogno di un mondo senza confini e di un'Italia meticcia, però questo non è il tempo e non è il luogo. Questo è il tempo e luogo in cui in Italia difende i propri confini. Questo è il tempo e luogo in cui l'Italia si dà delle regole sul tema dell'immigrazione, regole che prima non aveva. Questo è il tempo e luogo del Governo Meloni, che rispetta il patto con gli elettori.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Zampa.

È evidente che in queste condizioni saltano tutte le prerogative per un esame appropriato da parte della nostra Assemblea.

Allora riprendiamo e proviamo a vedere se va meglio. Sono altresì azzerate le prerogative dei senatori, che sono attribuite dall'articolo 72 della Costituzione e dovrebbero interessare anche alla maggioranza. Questa violazione è particolarmente grave

un giorno cambiare le forze, dovrebbe interessare il fatto che si calpesta continuamente il ruolo dell'opposizione e che questo Governo si sta specializzando in questa materia. È una violazione particolarmente grave nei confronti dell'opposizione, che viene privata di qualsiasi potere emendativo in ordine a un atto che ha forza di legge; questa violazione si ripete quotidianamente e ogni volta con fattispecie normative più discutibili. In questo decreto-legge è stato fatto confluire - è stato ricordato più volte, ma vale la pena ripeterlo - il decreto-legge n. 158, incamminato su un binario morto proprio qui nella nostra Assemblea. Assemblea. Voglio sollevare dubbi sull'esistenza delle condizioni straordinarie di necessità e urgenza, checché se ne sia detto poco fa, previste in maniera rigorosa dall'articolo 77 della Costituzione. Poiché chi mi ha preceduta dovrebbe avere studiato giurisprudenza, gli voglio raccomandare di andare a consultare e provare a rileggere cosa dice l'articolo 77 della Costituzione al riguardo. Queste condizioni mancano certamente e non sono state adeguatamente motivate con riferimento all'emendamento di cui al punto 6. Mi permetto anche di rinviare per altri delicatissimi rilievi alle considerazioni contenute nel parere del nostro Comitato per la legislazione e credo che sarebbe bene che i senatori andassero a leggere che cosa scrive il Comitato per la legislazione del Senato in un parere che è stato approvato nei giorni scorsi. Voglio anche soffermarmi sul fatto che il decreto-legge n. 158 è stato sostanzialmente prima emanato dal Presidente della Repubblica, poi derubricato a semplice emendamento e a voi questo è sembrato uno scherzo, mi sembra di avere capito dall'intervento che ho ascoltato. Il testo è stato manipolato, con la sostituzione delle sezioni specializzate dei tribunali con le ingolfatissime corti di appello, che vi hanno chiesto in tutti i modi di non procedere in questa direzione, e successivamente rispedito in Commissione per rispondere ai rilievi preoccupati che sono arrivati dal Quirinale e anche questo vi è sembrato uno scherzo, evidentemente. Questa intollerabile degenerazione della decretazione d'urgenza - non posso dimenticare le urla e gli strepiti che sentivo

e in questo caso evidentemente di noi senatori. Aggiungo a questo che un'ulteriore lesione recata all'effettiva partecipazione dei parlamentari alla decisione, riguarda anche l'esercizio del libero mandato ricevuto dai cittadini, che finisce in ultima analisi per ledere anche i diritti di questi ultimi. Ho fatto queste premesse per annunciare che, per questa ragione, proprio basandomi su una enunciazione della Corte costituzionale prospettata tempo addietro, comunico che, d'intesa con altri colleghi, in particolare la senatrice Camusso e il senatore Delrio,

daremo seguito a questo proposito. Vengo a questo punto ad alcuni contenuti di questo provvedimento. Ho già detto che è un ennesimo decreto e che questo davvero

un argomento che si può usare, né su cui si può sperare di contare, vi avverto anche che con quello che sta succedendo in Siria, come ormai denuncia qualunque quotidiano, se qualcuno di voi avesse la pazienza di leggerlo, lascia prevedere un arrivo molto importante di nuovi flussi migratori.

semina di odio e di paura presso i cittadini italiani. Si costruisce la paura del diverso, del migrante, diffondendo odio; ne sono una prova le eclatanti esternazioni di Vittorio Feltri, che nei giorni scorsi, giustamente - espressione di una maggioranza che si alimenta, alimenta e diffonde l'odio anti-migrante nel nostro Paese - hanno raggiunto un incredibile volgarità e violenza. Stupisce persino che si possa arrivare a tanto e che su questo tanto non si siano sentiti i pronunciamenti di alto livello, che sarebbero dovuti arrivare. Evidentemente si spera in questo modo di raccogliere voti presso gli italiani, ma, per nostra fortuna, possiamo anche dire che qualche sconfitta comincia a venire avanti e che probabilmente vi dovrebbe suggerire di cambiare strada. Dai vostri decreti-legge, dalle parole, anzi dagli *slogan* che voi utilizzate, emerge la chiara volontà di non affrontare il problema della migrazione e i problemi ad essa legati. La migrazione è un fenomeno molto complesso che ha bisogno di essere conosciuto, analizzato e accompagnato da provvedimenti utili se davvero si vuole spiegare ai cittadini che si sta facendo qualcosa. Non solo non vengono non vengono affrontati i problemi, ma tantomeno vi vediamo proporre qualche soluzione, come per esempio ha fatto la Spagna proprio nei giorni scorsi. Visto che sono state invocate altre espressioni del socialismo europeo che ci darebbero torto, guarda caso la Spagna ha fatto esattamente il contrario di quello che è stato detto.

descrivendo esattamente la *via crucis* che oggi, però, è molto peggio, per come voi l'avete costruita, persino di quella che allora hanno vissuto i nostri italiani. Se si vuole davvero provare a dare una soluzione e soprattutto a lavorare per la sicurezza e per la costruzione di una comunità più sicura e più solidale, queste persone hanno bisogno prima di tutto di emergere e di poter vivere un processo di regolarizzazione che va nella direzione opposta alla vostra. Avete fatto di tutto per non integrare; avete cancellato norme sull'accoglienza che avevano dimostrato di funzionare, funzionare, avete ripristinato i decreti Salvini e tolto la protezione speciale. Tutto questo lo fate nonostante che in tanta parte di questo Paese la società civile organizzata, il volontariato e le associazioni, in *partnership* con le amministrazioni pubbliche e le Istituzioni, in collaborazione e in cooperazione, abbiano saputo costruire - e quando le si va a vedere, si resta stupiti - buone prassi, esperienze positive che dimostrano che c'è una strada per costruire una soluzione al problema: trasformarlo addirittura in opportunità e in maggiore sicurezza. Tutto il decreto-legge è attraversato invece da una ideologia anti-migratoria. Voi ristabilite l'obbligo del migrante a collaborare, per esempio, per l'accertamento della sua identità; ottima cosa, peccato che decretiate la licenza di ispezione dei dispositivi elettronici anche delle persone minorenni e anche questo senza autorizzazione giudiziaria. Evidentemente avete molta paura di passare dai tribunali con le vostre e di confrontarvi con uno Stato di diritto che rispetta le persone anche, anzi soprattutto, nella loro condizione di maggiore fragilità fragilità data dal fatto che sono migranti. In questo modo violate l'articolo 13 della Costituzione. Parlate di sicurezza, ma appunto non regolarizzate quanti sono già qui e non gli date il tempo necessario a cercare un lavoro, facendoli finire così nella irregolarità. Concludo, Presidente, ricordando semplicemente un dato. Confindustria ci ha detto di avere bisogno di 100.000 nuovi ingressi, da finalizzare all'occupazione in settori cruciali come l'agricoltura e il turismo. E guardate che, con la crisi del settore manifatturiero, credo che provare a investire davvero sui comparti dell'agricoltura e del turismo sia una cosa importante. Bene, voi ne autorizzate 10.000 in via sperimentale per assistere anziani e disabili (10.000 contro i 100.000 che vengono chiesti dalla Confindustria) e avete stabilito, qui sfiorando davvero, secondo me, la crudeltà da un lato e, se mi è permesso, la stupidità normativa dall'altro, che i ricongiungimenti familiari debbano attendere il doppio di quello che è previsto oggi: due anni e non più uno; due anni di permanenza continuativa di uno dei componenti della famiglia. Raddoppiando i tempi, voi violate e ignorate tutti gli studi sul fenomeno migratorio, che ci dicono che la presenza della famiglia è un fattore importantissimo di stabilizzazione, che aumenta la sicurezza e il desiderio e la volontà di integrarsi. *(Applausi)*. Quindi passate da un errore all'altro, a dimostrazione del fatto che non volete assolutamente trovare una soluzione, perché pensate che questa sia una bandiera per tirare a casa qualche voto. E non lo avrete. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel dibattito avvenuto in Aula abbiamo sentito molte speculazioni e molte interpretazioni per così dire confuse su alcune parti di questo testo e, in generale, sull'approccio del Governo Meloni alla materia dell'immigrazione e soprattutto un sostanziale irrigidimento da parte delle opposizioni su prese di posizione puramente ideologiche, distanti dalla realtà e che non giovano né a risolvere il problema degli immigrati irregolari, né evidentemente quello della necessaria e indiscutibile tutela delle persone, tutela lapalissianamente mancata in tutti questi anni e che ha regalato al Mediterraneo il triste primato di fossa comune più grande e tragica della storia contemporanea. La superficialità e il buonismo imperanti nei precedenti Governi hanno lasciato problemi irrisolti ancora più grandi, come quello delle sacche di illegalità, ovviamente organizzate, che approfittavano e aggiravano le norme per usufruire a proprio vantaggio dei flussi migratori e restituire, come dato di confronto ad esempio in molti territori, solo il 3 per cento di contratti di lavoro rispetto al numero di persone in ingresso. Storture alle quali Giorgia Meloni ha voluto prontamente rispondere con una denuncia al procuratore nazionale antimafia, consentendo così un'accelerazione che ha portato a decine di arresti e a smascherare un meccanismo truffaldino consolidato da tempo e perpetrato sbeffeggiando le nostre leggi e i canali regolari. Superficialità e buonismo dei quali ha beneficiato la criminalità organizzata; ne cito una per tutte, la mafia nigeriana, che si è avvantaggiata proprio dei flussi migratori irregolari, consolidandosi sull'intero territorio nazionale. Questa è crudeltà. E allora voglio utilizzare il dibattito di oggi per porre un po' di ordine in tutto questo rincorrersi di dichiarazioni roboanti contro l'operato del nostro Governo e per evidenziare l'approccio di sostegno agli stessi migranti che fin qua è stato taciuto, suppongo con l'evidente volontà di disegnare un Esecutivo sempre pronto alla caccia dello straniero, mai solidale con le donne, con gli uomini e con i bambini (persone, nostri fratelli). Non potevamo, non possiamo credere di sconfiggere la tratta di esseri umani e le morti in mare facendoci le foto nei palazzi del potere con gli stivali sporchi di fango, per poi invocare il diritto alla moda e all'eleganza e scoprire di avere tra i propri familiari chi viene coinvolto in indagini su speculazioni con il *business* dell'accoglienza. Non possiamo credere che si possa gestire la più grande truffa ai sogni di migliaia di persone, che può costare anche 20.000 euro a viaggio, senza sicurezza dei mezzi con i quali effettuarlo e soprattutto senza certezza di arrivare sani e salvi a destinazione, semplicemente spalancando le frontiere d'Italia e d'Europa. Non possiamo chiudere gli occhi e non vedere che molte di queste persone, spinte dal desiderio di costruirsi un destino migliore, verranno presto private dei loro diritti esattamente da chi aveva loro promesso, per così dire, l'America, e nel nostro caso l'Italia, e che invece poi li trasformerà facilmente in manovalanza per criminali e sfruttatori. Non possiamo quindi prescindere da una regolamentazione efficace e strutturata, se vogliamo e dobbiamo perseguire un'accoglienza dignitosa e una integrazione concreta e duratura di queste persone. Cominciamo quindi dalla parte delle tutele, perché finora sui *social* e nei dibattiti su giornali e TV non ho sentito sottolineare che in questo provvedimento, ad esempio, sono previste delle misure a protezione dei lavoratori vittime di caporalato; non ho sentito spiegare che è stata introdotta, grazie anche a un intervento di Fratelli d'Italia, una quota fino al 40 per cento riservata alle donne nei settori del lavoro sociosanitario, e che è arrivata anche una proroga di sessanta giorni per utilizzare i nulla osta lavorativi scaduti, cominciando con una sperimentazione di 10.000 ingressi per il prossimo anno, da assegnare ad anziani e disabili.

sui ricongiungimenti familiari, e allora spieghiamolo una volta per tutte: la norma non si applica a chi ha diritto alla protezione internazionale, ed anzi noi con questo testo ne rafforziamo il principio, ribadendo che chi ne usufruisce deve essere visto come priorità rispetto ad altri. Da molti, poi, ho sentito preoccupazione rispetto alla tutela della *privacy* nel caso in cui si debba ricorrere a verifiche sui cellulari per consentire l'identificazione dello straniero e la ricostruzione della sua identità; preoccupazione più che lecita, ma che può essere cancellata dal fatto che da queste ispezioni rimangono precluse la corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione, il tutto quindi in piena conformità alle norme previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta di Nizza per quanto attiene alla protezione dei diritti dei dati di carattere personale e, non da ultimo, ai nostri princìpi costituzionali. Si è detto poi che l'Italia va contro l'Europa. Peccato che, ad esempio, questo testo sia anticipatorio del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, previsto dal regolamento UE n. 1348 del 2024, la cui entrata in vigore avverrà entro giugno 2026. Il nuovo regolamento stabilirà un procedimento comune di protezione internazionale dell'Unione, rendendo obbligatorie le procedure accelerate di frontiera, e prevedendo criteri più specifici rispetto alla definizione di Paese sicuro, che sarà legata al numero di domande di asilo in totale accolte dall'intera Questo con buona pace di chi ancora si interroga se sia lecito avvalersi della specifica di "Paese sicuro" per gestire i flussi e magari usare questi dubbi per bloccare, di fatto, i rimpatri, che sono indispensabili, improrogabili, indiscutibili, se si vuole perseguire l'obiettivo di una migrazione integrata e finalizzata a dare un secondo destino a chi sfida la sorte per crearsi una nuova vita in Italia. Perciò il tema non può essere che con questo testo si trasferisce alle corti di appello la competenza sulla convalida dei trattenimenti: intanto la competenza ad un giudice superiore non arretra, ma rafforza l'intervento in materia di diritti umani e civili. Il tema è se noi vogliamo continuare a far gestire il fenomeno delle migrazioni al caso, troppe volte al caos e in stato di emergenza, e sicuramente dai trafficanti di esseri umani e dalla criminalità organizzata. Il tema è se noi vogliamo che siano le ONG, quindi organizzazioni private con interessi privati, a decidere chi sbarca sul nostro territorio, dove sbarca, con quali tempi e secondo quali norme di diritto. Il tema è se vogliamo continuare a consentire che l'autorità giudiziaria, violando il principio della separazione dei poteri e del loro equilibrio, esprima valutazioni politiche nei provvedimenti giurisdizionali, oppure se queste competenze, come è giusto che sia, debbano tornare allo Stato e nello specifico al Governo e al Parlamento, che si assumono la responsabilità di provare a creare una strategia non solo locale di gestione del flusso migratorio, ma anche attraverso ragionamenti allargati ad un consesso europeo e ad una più stretta cooperazione internazionale. Anche per questo il Governo Meloni ha voluto istituire un tavolo tecnico per monitorare l'applicazione dei decreti flussi, per capire le anomalie e correggere le storture. Ha scelto di produrre un'informativa annuale sui Paesi sicuri mediante una relazione trasmessa alle Commissioni parlamentari per aggiornare, se necessario, quell'elenco in tempi consoni agli scenari politici. Ancora, ha voluto investire - si tratta di un investimento - il 7 per cento delle spese connesse all'accoglienza con il progetto Albania per una soluzione condivisa responsabilmente con un altro Stato. un caso di studio a cui vogliono guardare - pensate un po' - con attenzione altri quindici Paesi europei. In conclusione, è vero che noi abbiamo un'ossessione oggi ce ne assumiamo convintamente, ancora una volta, l'impegno. Questa ossessione è quella di affrontare il tema delle migrazioni, conciliando regole e diritti in nome della sicurezza e della dignità di tutti.

è un tema estremamente importante e fondamentale che caratterizza il nostro tempo ed è un tema che noi dovremmo - credo - approcciare con grande lucidità e freddezza, che è esattamente quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Voglio anticipare un'obiezione che ci viene sempre fatta: mi viene fatta quando parlo di questa questione pubblicamente, ma anche in sede privata, con amici o conoscenti. Mi chiedono perché questa cosa allora non l'abbiamo fatta noi. A parte il fatto che le maggioranze in questi anni sono state molto varie, ma in realtà quello che credo ha bloccato il Paese - e non soltanto il nostro, attenzione dal prendere una decisione razionale è stato l'incredibile surriscaldamento del dibattito pubblico su questa vicenda, una vicenda che avrebbe dovuto essere considerata di interesse nazionale, come una risorsa. una bruttissima espressione nelle aziende si parla del personale come "risorse umane"; a me non piace molto, anche se vengo da quel mestiere, però certamente l'intelligenza e il talento sono un elemento fondamentale della prosperità dei Paesi. Noi italiani ci troviamo, come altri tanti altri Paesi del mondo ricco, in una situazione abbastanza paradossale, che è quella di vivere una condizione demografica insostenibile. Lo sappiamo: abbiamo perso 200.000 nascite nel giro di quindici anni, che sono un numero enorme. Siamo passati da circa 560.000 a circa 360.000 nati dal 2009 al 2024. Questa mancanza di italiani che nascono nel nostro Paese è un problema da tutti i punti di vista: pensate semplicemente al pagare le pensioni, pensate pensate a tutte quelle persone che ci servono a portare avanti la pubblica amministrazione, la polizia, gli insegnanti, i medici, gli infermieri. già detto qualche minuto fa, durante la precedente discussione, che il Ministro della salute è andato a chiedere 10.000 infermieri al Ministro della sanità dell'India. Quindi, se il Ministro della salute italiano si rende conto che ha bisogno di chiedere all'India 10.000 infermieri è perché abbiamo oggettivamente un problema. Quindi, che cosa dovrebbe fare un Paese responsabile? Credo che dovrebbe sedersi a un tavolo e dire che abbiamo un problema di di scarsità di risorse umane, scarsità di talento, scarsità di intelligenze, di braccia e di teste, ma abbiamo una formidabile richiesta da parte di altri Paesi di persone che vogliono venire a prestarsi come braccia, come teste, come intelligenze e come talento. Quindi, dovremmo fare quell'operazione economica di incontro della domanda e dell'offerta, che andrebbe fatta con una logica molto fredda e razionale: dovremmo dire di quante persone abbiamo bisogno,

davanti a un fenomeno che andrebbe analizzato e risolto. Diciamoci una cosa, sottosegretaria Ferro: che la legge Bossi-Fini non sia stata cambiata

perché c'è una richiesta fortissima, da parte delle imprese e del Paese, di queste persone) ma, secondo la legge Bossi-Fini, le persone che vengono regolarmente in Italia non ci dovrebbero essere. In altre dovremmo avere un'offerta di lavoro fatta a una persona che vive in Senegal o Ecuador mai vista prima e dimostrare che non c'è una persona italiana che può fare quel lavoro. Mandiamo quindi il permesso di lavoro quindi il permesso di lavoro all'ambasciata italiana in Ecuador o Senegal e la persona arriva in Italia. Non funziona così, perché è ovvio che nessuno offre un lavoro a chi non

Anzitutto, sottosegretaria Ferro, se una persona straniera si trova in Italia e ha un contratto di lavoro, è in grado di spiegarmi in modo razionale per quale motivo debba essere un irregolare?

poi cose come questa vicenda dei centri in Albania, che veramente - mi permetta di dirglielo, Sottosegretaria - grida vendetta. Spieghiamo anche questo. A cosa servono questi centri in Albania? Servono semplicemente a dire che se tu vieni da un Paese sicuro, quindi la procedura di riconoscimento dell'asilo

Gli albanesi non vogliono le persone che sono nel centro. Pertanto, le tratteniamo lì per fare questo esame e poi le rimandiamo indietro dall'Italia.

non possono vivere o spostarsi in Albania, ma devono poi tornare in Italia. Anche la stessa causa per accertare il diritto all'asilo deve essere fatta in Italia. Spendiamo tutti questi soldi, utilizzando un miliardo Penso alla Polizia penitenziaria, di cui abbiamo bisogno come il pane. Siamo arrivati a 83 suicidi nelle carceri italiane, stiamo sfiorando il *record* assoluto. Siamo senza Polizia penitenziaria, ma abbiamo poliziotti penitenziari e Polizia

soltanto un'idea propagandistica: si vuole lucrare sulla paura, sulla preoccupazione e sulla diffidenza verso chi è diverso da noi. Noi, invece, dovremmo investire in formazione e coinvolgere in uno sforzo incredibile anche le aziende private, per poter utilizzare tutto questo talento in modo razionale. Signor Sottosegretario, io non penso che debbano entrare tutti, ma che il fenomeno debba essere gestito in modo più razionale. Che questa sia propaganda, poi, è dimostrato dal fatto che ci sono norme che si accaniscono contro le persone, perché si vuole dare un'idea muscolare.

per una classe dirigente responsabile di governare un Paese in questa epoca storica. Credo che stiate davvero abdicando alla vostra funzione di governare il Paese per dedicarvi a un'attività propagandistica che non fa bene a nessuno: forse a voi, ma comincio a dubitarne. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi scriviamo una pagina importante per il futuro del nostro Paese. Con l'approvazione del decreto flussi, diciamo basta alle promesse irrealizzabili e al caos che per anni ha segnato la gestione dell'immigrazione. Nel decreto non solo vengono maggiormente regolamentate le disposizioni in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, ma si pongono maggiori tutele ed assistenza anche alle vittime del caporalato. Questo decreto è una risposta concreta e coraggiosa, che nasce da un lavoro di squadra tra i territori e il Governo. Riprendendo un mio disegno di legge, il n. 502 del 2023, la stretta sui ricongiungimenti familiari, fortemente voluta dalla Lega, in particolare di quella del Friuli Venezia Giulia, di cui ho l'onore di essere segretario regionale, ne è l'esempio perfetto. Si tratta di una misura che non nasce a tavolino, ad opera di qualche burocrate rinchiuso nel palazzo, ma dall'ascolto diretto delle comunità, da quel rapporto stretto e continuo di chi vive i problemi quotidiani dei territori e ha il dovere di tradurli in soluzioni. La Lega è questo: un partito che parte dall'ascolto dei cittadini e porta le loro istanze fino a Roma. Siamo e continueremo ad essere una sentinella delle necessità locali, capace di trasformarle in politiche nazionali efficaci.

ma è applicata in molti altri Stati, tra cui la Francia del vostro mito, quel famoso Macron. Questa legge rivede i legge rivede i tempi per ottenere il ricongiungimento familiare, che saranno evidentemente più lunghi, permettendo di verificare con maggiore attenzione la stabilità della permanenza in Italia di chi presenta la domanda. Inoltre, sarà obbligatorio - altro passaggio importantissimo - dimostrare la conformità della struttura abitativa, perché i controlli finalmente diventeranno più stringenti. Non saranno più sufficienti dichiarazioni ed autocertificazioni vaghe e generiche, ma dovrà essere garantito che le condizioni di vita rispettino *standard* che, per noi, devono essere anche dignitosi. Questa misura non è solo una questione di ordine e di sostenibilità. È anche un atto rispettoso verso chi arriva, ma anche verso le comunità che accolgono. Con il decreto-legge in esame, unitamente a quanto proposto nella prossima manovra di bilancio in approvazione alla Camera dei deputati,

nella giusta direzione. È una scelta di responsabilità, ma anche di giustizia sociale, che tutela le risorse degli italiani, in un momento storico come quello attuale, quando ogni euro deve essere speso per rispondere alle vere priorità di questo Paese: il sostegno alle famiglie, il rafforzamento dei servizi essenziali e la crescita economica. Non si può più accettare che chi lavora e paga le tasse in Italia debba vedere le proprie risorse disperse in meccanismi poco controllabili e spesso abusati. Permettetemi allora di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato. Desidero in particolare ringraziare il sottosegretario Molteni, esempio di dedizione e competenza, ma anche tutta la squadra della Lega, che ha lavorato con determinazione per trasformare le richieste dei territori in norme chiare e incisive. cari colleghi, è il nostro modo di fare politica: ascoltare, agire e poi portare a casa risultati. A differenza di chi, in passato, ha scelto la strada dell'immigrazione incontrollata e delle porte aperte senza alcuna responsabilità, noi vogliamo invece mettere ordine. La sinistra ha illuso i migranti, li ha trattati con un sistema incapace di garantire loro un futuro dignitoso, scaricando costi e problemi sulle spalle degli italiani e delle nostre comunità. Per citare proprio il sottosegretario Molteni, disumano non è chiedere regole e rispetto; disumano è continuare a perpetuare questa illusione, prospettando ai migranti opportunità che non ci sono e che non possono essere garantite. Il decreto-legge flussi, quindi, non è solamente una legge, è un segnale davvero di svolta; è la dimostrazione che, con un lavoro di squadra tra territori e istituzioni, si possono affrontare davvero e risolvere questioni complesse come quella migratoria. È la prova che la politica può tornare ad essere vicina ai cittadini, attenta alle loro esigenze e pronta a risposte con azioni concrete. Concludo il mio intervento, di chi sa che oggi non stiamo solo cambiando le regole, ma stiamo costruendo un'Italia più forte, più giusta e più rispettosa soprattutto delle sue comunità e dei suoi cittadini; un'Italia che sa guardare al futuro con responsabilità e determinazione.

Come al solito, vi siete ridotti all'ultimo minuto, contraendo il dialogo democratico. Ve lo dico io perché succede questo: Ve lo dico io perché succede questo: quando si parla di immigrazione, vi scatta una molla, entrate in *tilt* e allora cominciate a essere presi dalla sindrome dell'iperproduzione normativa. Quando fate questa scelta di normare e di rimaneggiare continuamente le vostre regole, combinate pasticci giuridicamente imbarazzanti. Avevate emanato un decreto-legge sui Paesi sicuri, su cui eravamo pronti a confrontarci in Commissione; poi però avete cambiato idea, perché vi siete resi conto che avreste dovuto affrontare un dialogo democratico, ma a voi il dialogo democratico non piace

A voi non piace neppure la Costituzione, perché vostro malgrado prevede qualcosa a cui sembra che siate un po' allergici, ovvero il bilanciamento dei poteri e lo Stato di diritto: voi non lo volete lo Stato di diritto; voi volete lo Stato di polizia, state varando un provvedimento sicurezza liberticida. Sul bilanciamento dei poteri cosa dire? Voi state facendo un premierato che è un sistema che sbilancia tutti gli equilibri che la Costituzione e i Padri costituenti avevano fissato per garantire la democrazia e la libertà dei cittadini.

è troppo difficile per voi riconoscere che il protocollo Italia - Albania è un clamoroso fallimento?

Veramente qui dimostrate di essere i maghi della manipolazione, capisco su cosa si basano i vostri consensi: sulla manipolazione o su promesse elettorali che poi non riuscite a realizzare perché erano irrealizzabili. Quello che davvero esonda qui sono i provvedimenti: siamo arrivati all'ottavo provvedimento, uno più inefficace dell'altro, perché non siete riusciti a dare una risposta univoca, dato che continuate con i decreti e non pensate che ci vorrebbe magari un solo disegno di legge, ma fatto bene. Qui state dimostrando un dilettantismo giuridico che fa paura. Se entriamo nel merito - e qui effettivamente entrare nel merito è un po' difficile, visto che non abbiamo avuto tempo di affrontare il tema in Commissione - state mostrando il peggio - state mostrando il peggio dell'arroganza legislativa. Ve la siete presa anche con misure punitive nei confronti della magistratura, perché non so spiegarmi altrimenti il taglio delle sezioni specializzate dei tribunali, che va a ingolfare poi le corti d'appello.

di Sharm El Sheik, perché non si può sentire. Voi state confondendo la sicurezza che viene garantita ai turisti che portano soldi con la sicurezza dei cittadini, perché in quel Paese chi si oppone al regime viene torturato e si finisce in carcere anche se si indossa una maglietta per protestare contro la tortura.

ma allora quali sono questi valori? Vale solo la vostra famiglia e quella degli altri non conta niente? A me sembra sempre più chiaro che questo Governo sappia solo fare propaganda, una propaganda muscolare, ma non sappia risolvere i problemi: sa soltanto alzare la voce e fare la voce grossa con le categorie più deboli, ma quando si tratta di colpire i colletti bianchi o combattere contro la corruzione, che ci costa più di 230 miliardi l'anno, allora lì cominciate a essere benevoli, cominciate a concedere benefici penitenziari anche a chi non vuole collaborare con la giustizia.

vi scatta la molla: avete questa ossessione dell'immigrazione in generale, ma non siete capaci di andare alle cause del problema. Dovete prima comprendere le ragioni per cui la gente

l'immigrazione, la prima cosa che dovete fare è essere contro la guerra e contro la vendita indiscriminata delle armi. *(Applausi)*. Il nostro Gruppo è contro la guerra, si vuole battere anche perché si facciano politiche per promuovere la pace, perché se continuate a soffiare sul fuoco e ad alimentare le guerre, allora siete i primi complici di un sistema che alimenta ed incrementa l'immigrazione. Signor Presidente, serve una politica intelligente. Se la politica riuscisse a comprendere queste cause, allora si dovrebbe rendere conto che è importante lavorare innanzitutto sull'integrazione, ma soprattutto sulla cooperazione internazionale, perché senza di essa sarà una battaglia persa. Sono queste le misure che risolvono il problema e possono arginarlo, non è il protocollo Italia-Albania. Le persone infatti smetteranno di fuggire dalle loro terre quando non ci sarà più bisogno di farlo. Voi però Voi però prendete la strada della propaganda e preferite parlare alla pancia degli italiani. Peccato però che finché continuate a fare propaganda, la gente continua a morire nelle sue terre e noi continuiamo a perdere tempo qui con i vostri provvedimenti che non servono a niente.

Voi avete una posizione ideologica ad esempio contro le ONG, che di solito fanno un lavoro che dovremmo tutti ringraziare, perché salvano delle vite,

che vuole. Le regole garantiscono la democrazia e il processo democratico. Vorrei fare invece un altro tipo di intervento: di merito, in questo caso. Mi chiedo e vi chiedo con l'inverno demografico che abbiamo nel nostro Paese, stiamo ancora discutendo di flussi migratori? Oppure invece dovremmo discutere

fame nel mondo, desertificazioni, guerre. Quelle sono guerre fatte dall'Occidente, ad esempio, in Medio Oriente oppure in Afghanistan, prima dall'Unione Sovietica e poi

magari con l'aereo e un permesso di soggiorno. Poi si parla di caporalato, ma, quando vengono qui, c'è qualcuno che deve dargli una mano. E chi gliela dà? Non lo Stato. Sono singole persone:

Nella bassa Lombardia e nell'alta Emilia nelle stalle ci sono i *sikh*, che non vengono con i barconi.

Il problema è: c'è un ufficio di collocamento che prepara quei lavoratori (immigrati e non) a fare questi lavori? Abbiamo un censimento di quelli che ci sono? No, lo Stato manca.

non c'è un italiano che fa questo lavoro. Vale anche per il Veneto, o no? E allora facciamo finta che questo non c'è?

questa è una responsabilità morale e politica *(Applausi)* che deve avere la comunità occidentale, prima di tutto. Quei ragazzi non hanno mai visto la pace nella loro vita, che non hanno mai potuto affrontare in modo diverso, ed hanno fatto due anni di cammino a piedi per arrivare nell'Occidente, ma noi li respingiamo, li mettiamo in galera o gli diamo le bastonate. Credo che questa non sia umanità, ma un modo per creare muri. Io invece sono per creare ponti e continuerò a farlo.

siamo all'ottavo provvedimento di questo Governo in materia di immigrazione e molti di questi provvedimenti in realtà sono contraddittori, si contraddicono l'un l'altro, o si superano tra di loro in propaganda. Presidente, siamo passati dal blocco navale, per capire ben presto che era una cosa irrealizzabile, alla caccia agli scafisti nel globo terracqueo, per poi capire che in realtà gli scafisti su quelle navi non ci salgono o, se ci salgono, sono i primi ad andare via e ad abbandonarle, fino a passare alla deportazione coatta in due centri in Albania che ci sono costati un miliardo di euro, con i viaggi più costosi di sempre: circa 250.000 per ogni viaggio della nave Libra, che ha portato di fatto poche decine di migranti in questi centri per poi riportarli in Italia. Tutto ciò dovrebbe far capire a questo Governo e a questa maggioranza che il fenomeno migratorio va governato, ma non può essere

per non parlare di tutte le persone che lasciano i loro luoghi d'origine per guerre, carestie e povertà. In realtà, sono anche i dati economici che ci dicono che questo fenomeno va governato. Basterebbe saper leggere, per esempio, le tabelle del dove c'è scritto chiaramente che, se non proviamo ad integrare la forza lavoro anche con quella che è rappresentata oggi dai migranti, noi avremo un calo del nostro PIL e quindi della crescita della della nostra economia. Purtroppo, però questa maggioranza continua non solo a voler fare propaganda, ma a distorcere la realtà e allora confonde il soccorso con l'accoglienza e cerca di trasmettere ai cittadini italiani l'idea che c'è un'invasione di migranti. signor Presidente, basterebbe guardare i dati: quest'anno 64.000, l'anno scorso 150.000, ma quanti sono i profughi ucraini che abbiamo accolto in un anno? Quasi 200.000. Abbiamo la percezione di essere invasi dagli ucraini? No, assolutamente no. Perché abbiamo invece la percezione di essere invasi dalle persone che arrivano dall'Africa o dal Medio Oriente? Perché c'è la volontà di demonizzare il migrante e di far percepire al cittadino italiano che le difficoltà drammatiche che stanno vivendo oggi i nostri cittadini sono dovute ai migranti, quando non è assolutamente così.

bocciate alla Camera, perché qui in Senato non abbiamo nemmeno avuto il tempo e il modo di discuterle. Avevamo chiesto, per esempio, di introdurre il permesso di lavoro, perché è fondamentale che il datore di lavoro conosca il lavoratore, ma anche questa proposta è stata bocciata per continuare a mantenere come unico criterio per il permesso di soggiorno il *click day*, che assolutamente non può essere la soluzione a quell'integrazione che invece noi chiediamo. Avevamo chiesto la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per fare anche altri lavori: chiaramente anche questo emendamento è stato bocciato. Avevamo chiesto di prevedere che ci potesse essere un garante, uno *sponsor,* per ottenere il rilascio del permesso. Avevamo chiesto di potenziare i ricongiungimenti familiari questo provvedimento è andato in direzione totalmente opposta. Sono diventati più difficili i ricongiungimenti familiari, perché oggi bisogna aspettare due anni: alla faccia del Governo che mette al primo posto la famiglia.

deriva dalle normative internazionali, che sono universali. È stata anche affidata direttamente ai questori la possibilità di sequestrare i dispositivi dei minori e poi, cosa per me più grave, è stata ulteriormente decapitata attività di ricerca e di soccorso in mare da parte delle navi ONG. È stata estesa anche agli armatori la responsabilità in caso di fermo di quelle navi ed è stata potenziata la fornitura di armi e motovedette ai Paesi terzi. Per non parlare dell'obbligo per gli aerei di supporto alle navi ONG di obbedire alle autorità libiche e tunisine: gli aerei di supporto, che sono quelli che hanno denunciato le barbarie della guardia costiera libica devono oggi obbedire agli ordini delle autorità libiche e tunisine. Sembra esserci veramente l'ossessione di impedire il soccorso. Presidente, non ho paura di dirlo: per me bloccare una nave che soccorre migranti in mare equivale a bloccare un'ambulanza, è esattamente la stessa cosa. *(Applausi)*. Il nostro Mediterraneo è diventato un cimitero. Ci sono 30.000 morti sul fondo del Mediterraneo, molti dei quali non hanno nemmeno un nome, perché non è previsto il riconoscimento sul DNA di quei cadaveri, che quindi non vengono restituiti alle famiglie neppure quando sono recuperati dal fondo del mare. Uso questo ultimo solo per porre all'attenzione di questo Governo un ultimo caso, sul quale chiaramente mi accingo a depositare un'interrogazione, quello della nave Geo Barents, che il 28 novembre, con a bordo un *team* di Medici senza frontiere, ha salvato 83 migranti, però da un barcone su cui ce n'erano più di 100. Sa cos'è successo, Presidente? Quando la nave si apprestava a raccogliere i migranti, sono arrivati due mezzi libici con a bordo uomini armati, che hanno sparato in aria per obbligare gli uomini a lanciarsi dal gommone e poi hanno sequestrato

quei mezzi libici, si è gettato in mare per provare a salvare la sua famiglia e non faceva altro che urlare: così continueranno a stuprarla! Perché nei *lager* libici, dove vengono rimpatriati e dove sono stati portati anche quelle donne e quei bambini, succede questo:

dobbiamo fare altro: dobbiamo lavorare in ambito europeo e superare il Paese di primo approdo e, quindi, il Regolamento di Dublino. Anche qui mi chiedo perché questa maggioranza ha votato contro la riforma di quel Regolamento che, invece, è l'unica cosa che veramente serve. La propaganda resta zero, soprattutto quando di mezzo ci sono le vite delle persone e l'umanità di cui ha parlato anche il senatore Magni.

problemi politici seri - il decreto flussi e gli ingressi regolari in questo Paese sono un problema politico serio che riguarda l'interesse nazionale - ma sempre mescola l'interesse nazionale e i problemi politici seri con problemi di propaganda. Purtroppo, da secoli, la più grande arma nelle mani della politica è la paura. Non c'è niente di più forte che evocare paura: la paura del diverso, la paura del lontano. Questo Governo non rinuncia mai a questo esercizio. Non vi rinuncia nemmeno oggi, al punto che, dopo otto decreti sull'immigrazione, la domanda che mi faccio - pur essendo sinceramente pronto alla discussione su come migliorare l'interesse nazionale, anche e soprattutto favorendo l'immigrazione regolare - è se, invece che una pregiudiziale - lo dico ai colleghi che hanno esposto così bene

si potrebbe togliere il telefonino? A un italiano dell'Argentina che chiede il ricongiungimento familiare si potrebbe dire no, aspetti di più? Stiamo facendo categorie tra persone? Stiamo dicendo che, sostanzialmente, esistono esseri umani di serie A e di serie B? Mi chiedo, signora rappresentante del Governo, conoscendo la sua sensibilità, se non stiamo costruendo una nuova categoria politica e giuridica del clandestino, perché ci serve. Ciò invece che concentrarci

L'ingresso non è possibile con gli attuali canali. Io pongo anche un altro problema alla rappresentante del Governo per suo tramite, signora Presidente. Attenzione, perché noi parliamo di irregolari, ma una persona che entra illegalmente in Italia non è irregolare, non è clandestina: una persona che entra illegalmente in Italia ha diritto, secondo le leggi internazionali, a essere a essere trattata come una cittadina in attesa che venga riconosciuto eventualmente il suo diritto alla protezione internazionale. Non è una clandestina. Attenzione, dopo due mesi può lavorare. lavorare. Se voi continuate a dire che chiunque è irregolarmente in Italia è un clandestino ed è un pericolo, state costruendo questo immaginario di cittadini di serie A e di serie B e quelle persone non hanno più diritto ad avere diritti. Il diritto di asilo è non una concessione, ma un valore universale che non può essere limitato nemmeno dalla sacralizzazione dei confini che voi state facendo. Voi state cercando di dire agli italiani che state rendendo sacri i confini. C'è un Ministro che addirittura dice di essere sotto processo perché ha difeso i confini. No, non è così. È sotto processo perché ha violato i diritti di una persona a sbarcare, come prevedono le convenzioni internazionali. *(Applausi)*. Io non tifo perché venga condannato, ma non facciamo confusione. La sacralizzazione dei confini non vi dà il diritto di annullare il diritto internazionale. Questo non vi è consentito, altrimenti torniamo al pericolo di uno Stato totalitario. Hannah Arendt è stata apolide per diversi anni. A un certo punto della sua della sua vita ottiene il passaporto americano, dopo che nel 1937 le leggi razziali lo avevano sospeso, e dice di avere il passaporto, il libro più bello che conosca. Avere il passaporto vuol dire sentirsi parte di una comunità. Queste persone hanno diritto di essere trattate come persone, al di là della sacralità della persona umana, che non potete mettere in discussione nemmeno con il nono decreto sull'immigrazione. Hanno diritto a essere trattate come persone e soprattutto il diritto ad essere trattate non come clandestini, perché non solo clandestini. Siccome - come lei sa - le commissioni giudicatrici in media, per il 50 per cento, accolgono le richieste di protezione, questo significa che almeno per la metà di queste persone vale quello che io sto dicendo.

Spero che abbiate mandato una lettera alla Presidenza della Camera e una lettera anche alla Presidenza del Consiglio, perché - come dice il Comitato per la legislazione, come dice una sentenza della Corte costituzionale, come dice il Presidente della Repubblica - quello che è stato fatto, cioè l'unione dei due decreti, è una cosa illegittima, è una cosa sbagliatissima, che non consente l'esercizio dei poteri parlamentari. Siamo anche ben pagati - diamo questa notizia - per farlo e non possiamo fare il nostro mestiere. Mi dovete spiegare perché, su un argomento così decisivo per il futuro dell'Italia, come il tema dell'immigrazione, così importante, così strutturale, così serio, dobbiamo correre, unendo due decreti e facendo un pasticcio che non ha precedenti nella storia repubblicana. Io spero di poter vedere una lettera di protesta. Posso garantire che, al vostro posto, io l'avrei già mandata e l'ho già fatto in altre occasioni, ricoprendo altri ruoli, perché questa cosa è inaccettabile. Noi abbiamo una teoria, che cercherò di illustrare nei pochi minuti che ho. La teoria riguarda l'approccio poliziesco e di ordine pubblico che state mettendo in campo sul problema dell'immigrazione, a parte qualche segnale

in tutta questa legislazione c'è un filo conduttore, ossia si trasformano in reato l'ingresso e il soggiorno irregolare. Quindi, spostiamo l'attenzione dal problema di governare un fenomeno, di favorire l'immigrazione regolare e di capire qual è l'interesse nazionale, per l'industria e per la società. Sappiamo che l'immigrazione, oltre a essere la più potente arma politica collegata alla paura, è anche la più potente arma di trasformazione delle società occidentali. Il Canada, il Brasile, gli Stati Uniti non si sono forse trasformati grazie all'immigrazione? Non è stato forse un clamoroso processo di trasformazione culturale e sociale? Non sono arrivate solo braccia: sono arrivate teste. Andate nei più grandi laboratori di ricerca degli Stati Uniti. Io ho avuto la fortuna di lavorare in uno di essi. In ogni stanza vi è un'etichetta con un nome e una provenienza diversa: stanza. Gli uomini sono così: sono meravigliosi, sono unici e questo non dipende da dove sono nati. Possono trasformare il mondo, anche essendo nati in Sudafrica o in Pakistan, perché sono unici. Pertanto, questo atteggiamento securitario, quasi etnocentrico, in cui bisogna per forza trasformare uno che perde il lavoro in un soggetto illegale, è un approccio perdente. Usatelo per la propaganda, ma non usatelo se volete parlare dell'Italia e del suo futuro.

gli danno un fogliettino con un appuntamento e, dopo un anno, gli danno un'altra cosa e noi impegniamo straordinari prefetti, poliziotti - a loro va il nostro ringraziamento - a fare cose che non dovrebbero fare, perché l'immigrazione non è un problema di ordine pubblico. Diamoci anche questa notizia: il problema di ordine pubblico è l'emarginazione; diventa un problema di ordine pubblico quando c'è l'irregolarità, perché non è vero che gli immigrati che lavorano delinquono più degli italiani. Dove lo avete letto? Dov'è scritto? Gli immigrati che lavorano, di solito, rispettano di più le leggi.

Io credo che noi dovremmo discutere di questo, degli ingressi irregolari, della capacità di mettersi a sedere, perché riguarderà chi governerà dopo. Noi abbiamo commesso molti errori, moltissimi. molti errori, moltissimi. Io li testimonio, sono pronto a farlo, ma lo vorrei fare in un'Aula del Parlamento, discutendo serenamente di cosa serve al mio Paese. Voi non state discutendo di cosa serve al nostro Paese. Addirittura vi dimenticate di una cosa, ovvero del fatto che la parola «integrazione» non è un costo. C'è stato un famoso filosofo che ha detto: quando qualcuno mi chiede o vi dice che la parola educazione è un costo, riflettete su quanto vi costerebbe l'ignoranza.

il decreto-legge che oggi siamo chiamati ad approvare non è un semplice decreto flussi che stabilisce quote precise per l'ingresso di lavoratori extracomunitari, ma è la dimostrazione del continuo impegno del Governo Meloni sia nella lotta contro l'immigrazione clandestina, sia nel garantire diritti e dignità a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro provenienza. Se, da un lato, questo decreto prevede controlli più efficaci sui flussi di immigrazione legale, al fine di evitare frodi ed irregolarità, come emerso dal monitoraggio e dal confronto tra ingressi per finalità lavorative e contratti di lavoro effettivamente sottoscritti (cosa che chiaramente ha fatto ipotizzare che i flussi per ragioni di lavoro siano stati utilizzati da gruppi criminali riusciti a infiltrarsi nella gestione delle domande come canale ulteriore di immigrazione irregolare,

dall'altro lato, prevede anche norme che mirano a combattere lo sfruttamento dei lavoratori e a garantire una maggiore tutela alle vittime che contribuiscono a far emergere il fenomeno del caporalato, tanto che chi collabora proficuamente avrà il diritto a permanere legalmente in Italia, a seguire un corso di formazione e ad essere inserito nel mondo del lavoro, innestandosi così in un tessuto economico Sempre poi nell'ottica di un'efficace gestione dei flussi, mi preme anche evidenziare che nel decreto è stata inclusa la lista dei Paesi sicuri per i rimpatri, che diventa così norma primaria. Fra l'altro, l'elenco è stato conformato alle indicazioni derivanti dalla sentenza della Corte europea del 4 ottobre scorso, in base alla quale sono stati espunti tre Paesi - Camerun, Columbia e Nigeria - che, nel precedente elenco, presentavano eccezioni di carattere territoriale. L'individuazione dei Paesi sicuri per i rimpatri è competenza degli Stati membri, come riaffermato anche dalla recente sentenza della Corte di giustizia; questo perché la direttiva europea che introduce le procedure accelerate di frontiera se, da un lato, stabilisce che uno dei requisiti per l'applicazione sia proprio che il migrante irregolare provenga da un Paese sicuro, dall'altro lato, non definisce alcuna lista dei Paesi sicuri, demandandola perciò alla competenza degli Stati membri. Ne consegue che interpretazioni diverse dalla sentenza della Corte europea - come è avvenuto potrebbero portare alla potenziale paralisi del meccanismo dei rimpatri, perché si potrebbe arrivare al paradosso di valutare insicuri la quasi totalità dei Paesi del mondo. Una soluzione per uscire da questo stallo, visto anche quello che sembrerebbe essere l'orientamento della Corte di cassazione, potrebbe essere l'anticipazione dell'entrata in vigore del Patto per la migrazione e l'asilo

tassello che ci consentirà di evitare morti in mare, di spezzare l'orrendo *business* della tratta degli uomini e di garantire all'Italia una gestione non emergenziale dei flussi.

Voglio ricordare temporalmente i provvedimenti e le azioni diplomatiche, partendo dai primi due decreti approvati dall'inizio del 2023, cioè il decreto sulle ONG, il decreto Cutro: il primo regolamenta il comportamento delle ONG nelle operazioni di ricerca e ricerca e soccorso e in particolare regolamenta la disciplina dei salvataggi multipli; il secondo contiene una stretta sui trafficanti con pene più severe, prevede la perseguibilità degli scafisti oltre i confini italiani e introduce procedure accelerate di frontiera per i migranti provenienti da Paesi sicuri. A seguire, voglio ricordare la firma a luglio 2023 del Memorandum d'intesa fra il Presidente della Tunisia e Von der Leyen, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio, per stabilizzare i Paesi in crisi economica e sociale, ma anche per fermare le partenze dei migranti; tanto che già a settembre del 2023 gli arrivi, che in agosto avevano toccato il picco più alto, erano diminuiti. A ottobre 2023, poi, col decreto flussi, abbiamo superato la logica della sanatoria *ex post* degli ingressi irregolari, tanto cara alla sinistra; abbiamo riformato i centri di permanenza per i rimpatri, stanziando anche fonti per realizzarne dei nuovi, e abbiamo approvato il decreto immigrazione, che introduce espulsioni più rapide e controlli più accurati sui minori non accompagnati. A novembre, invece, è stato firmato l'Accordo Italia-Albania per la creazione di due strutture a giurisdizione italiana per la gestione delle domande d'asilo e dei rimpatri dei migranti soccorsi in mare; accordo che molti Stati europei - piaccia o no alla sinistra nostrana - stanno guardando con interesse, per non dire ammirazione, e che ha già avuto un chiaro effetto deterrente. È significativo infatti l'aumento del numero dei migranti che, quando arrivano, presentano un documento di identità: cosa che consente l'immediata identificazione non solo delle persone, ma soprattutto dei Paesi di provenienza. Fino a poco tempo fa, la maggior parte arrivava in Italia senza documenti. Con questo Accordo, per tanti aspetti - lo si voglia ammettere o no, comunque inaugurerà una fase completamente nuova nella gestione del problema migratorio - si realizza una delle tante proposte di Fratelli d'Italia che prevede la creazione di *hotspot* nei Paesi extraeuropei, proprio per valutare le richieste d'asilo e determinare, a monte, Prima ho ascoltato la collega Maiorino che ha sostenuto che, per le strutture in Albania si sprecano i soldi degli italiani. Non mi sembrava altrettanto preoccupata quando invece si sprecavano veramente per il superbonus, i banchi a rotelle che adesso sono finiti al al macero, i monopattini e altre amenità. *(Applausi)*. Detto questo continuo nell'elencazione. A gennaio 2024 si è svolta a Roma la Conferenza Italia-Africa, con cui è stato avviato il Piano Mattei, dando vita ad una nuova stagione di cooperazione con il Continente africano. Questo perché il Governo Meloni che - come dicevo prima - ha una strategia ben precisa e cerca soluzioni strutturali e non di facciata, vuole sradicare le motivazioni che spingono tanti africani a migrare, creando condizioni di sviluppo che consentiranno a noi di ottenere sostegno sia in tema energetico che in tema migratorio, e agli africani garantiranno quello che Papa Benedetto chiamava il diritto a non migrare. È sempre merito di Giorgia Meloni se oggi la maggioranza delle Nazioni europee segue la linea italiana sull'immigrazione. Sin dal suo insediamento, infatti, il Governo Meloni ha posto il tema migratorio nei principali consessi internazionali, dai Consigli europei ai vertici G7, da ultimo quello svoltosi in Italia, dove il tema ha trovato ampio spazio nelle conclusioni. Lo stesso patto per la migrazione e l'asilo, che citavo prima, di aprile scorso, recepisce proprio l'impostazione portata avanti dal Governo italiano e, cioè, asilo e protezione a chi ne ha diritto, difesa e controllo delle frontiere esterne dei flussi irregolari e lotta ai trafficanti e agli scafisti. Non possiamo più permetterci di gestire i flussi migratori in modo improvvisato o ideologico, e il cambio di passo rispetto ai precedenti Governi è evidente, non solo per la riduzione degli arrivi, ma soprattutto nel calo dei morti e dispersi in mare. Non avremo più un'immigrazione incontrollata, perché non si permetterà più che le quote di immigrati irregolari vadano ad esaurire la capacità di ricezione dell'Italia, come è stato fatto negli ultimi anni. Questo decreto-legge ribadisce infatti la volontà del Governo di creare le condizioni per permettere l'arrivo di migranti irregolari, evitando però truffe e infiltrazioni di gruppi criminali nei meccanismi di ingresso legali, ma soprattutto evitando quanto fatto negli anni precedenti, e cioè un'accoglienza indiscriminata e ideologica, penalizzante non solo per l'Italia ma anche per gli stessi immigrati, dovuta all'incapacità dei Governi precedenti di avere una visione strategica e lungimirante di un fenomeno di dimensioni mondiali. Una visione strategica che invece questo Governo possiede, come dimostrano tutte le azioni diplomatiche e tutti i provvedimenti che ho elencato. E la possiede perché è convinto che l'immigrazione irregolare debba essere combattuta in modo strutturale e che i flussi debbano essere gestiti dai Governi legittimamente eletti e non certo dai trafficanti, dagli scafisti o dai gruppi criminali, come è emerso dei controlli sulla gestione dei *click day*. *(Applausi)*. Mai era stato fatto tanto sul tema dell'immigrazione ed è indubbio che tutto questo impegno stia dando i suoi frutti; pur di colpire un Governo non gradito, pur di nascondere la propria incapacità di fare proposte costruttive, è disposto a danneggiare e screditare l'Italia intera, arrivando addirittura a chiedere all'Europa una procedura di infrazione su un provvedimento approvato dal Parlamento italiano solo perché non lo condivide. Che dire Presidente? Dei veri patrioti.

reiterato negli anni, svolgono un ruolo prezioso e impagabile nel far crescere eticamente e culturalmente la loro comunità e, quindi, il Paese stesso. Germano Cis, classe 1940, era una di queste persone. Nel suo paese, Bezzecca in Val di Ledro, quella della battaglia di Garibaldi e del famoso "obbedisco!", un parroco lungimirante pensò e realizzò, grazie alla donazione di una famiglia benestante locale, un cinema parrocchiale, sull'esempio di altri che nacquero in quegli anni nelle vallate alpine (altri due nella sola Val di Ledro). Era il cinema Don Bosco, nel 1948. Fin da bambino Germano fu affascinato dal cinematografo. Trascorreva al Don Bosco ogni momento libero; imparò presto i trucchi del mestiere e a quattordici anni, nel 1954, fu promosso proiezionista. Accanto al proiettore teneva sempre un sacco di sabbia e una coperta, da usare in caso di incendio; le pellicole erano allora altamente infiammabili. Lo fece per quarantaquattro anni, fino alla chiusura del Don Bosco nel 1998. Germano lavorava nella famiglia cooperativa, l'unico negozio di alimentari del Paese, di cui divenne direttore, e inoltre faceva il sacrestano in parrocchia e gestiva il cinema con il paziente sostegno della moglie Giacomina. Si era creato con il tempo una rete di contatti con l'ambiente cinematografico, che gli consentivano di intercettare le pizze dei nuovi film che approdavano in Italia lungo l'asse del Brennero. Concordava un appuntamento con le case di distribuzione e, al momento opportuno, partiva in auto da Bezzecca per recarsi al luogo concordato per la consegna, talvolta fino a Padova, dove esse avevano sede. Sceglieva i film da proiettare con l'assenso del parroco e ne prendeva in consegna le pizze, che restituiva qualche settimana dopo nello stesso modo. Negli inverni lunghi e freddi della Val di Ledro, allora pressoché isolata e povera di offerte culturali, il cinema Don Bosco offriva alla gioventù del luogo le poche occasioni di aggregazione, di intrattenimento e di apertura al mondo. La sala era riscaldata con la stufa a legna e non di rado i ragazzi portavano con sé qualche fascina, che sostituiva i soldi per il biglietto. Nella piccola sala arrivarono a stiparsi fino a 300 persone, usando appositi strapuntini. Non c'erano ancora le norme sulla sicurezza dei locali, ma per fortuna non ci furono mai incidenti. Va da sé che, quando nel 1988 uscì il film "Nuovo cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore, questo piacque particolarmente a Germano, che lo riguardò molte volte, rivedendo sé stesso nei panni del proiezionista Alfredo. Oggi il cinema Don Bosco non c'è più e al suo posto c'è il nuovo centro culturale del Paese, frequentato più dagli anziani che dai giovani. Ma così va il mondo. Germano Cis ci ha lasciati il 27 novembre. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Bezzecca, a pochi metri dalla chiesa, dal negozio e dall'area dove sorgeva il cinema Don Bosco: i luoghi della sua vita e della sua comunità, che ne conserverà a lungo la memoria. *(Applausi)*.

Io appartengo a una delle generazioni che è cresciuta con la paura anche del contagio. Oggi invece non si parla più di AIDS, eppure ogni anno i nuovi contagi nel mondo sono un milione e mezzo. I contagi sono in aumento, soprattutto da dopo la pandemia, anche in Italia. L'ultimo *report* recentissimo dell'Istituto superiore di sanità, di novembre 2024, ha evidenziato una ripresa dei contagi da HIV soprattutto nella fascia adolescenziale, nei ragazzi tra i anni. Questo avviene, Presidente, anche perché si parla troppo poco di HIV: non c'è formazione, non c'è informazione, non c'è prevenzione. Eppure, oggi esistono addirittura dei test rapidi per la diagnosi da HIV, dei test salivari che abbiamo presentato oggi in una conferenza qui in Senato. In questi anni In questi anni moltissimo ha fatto la ricerca per individuare nuovi metodi di diagnosi, ma anche nuove terapie che permettono alle persone contagiate dal virus HIV di convivere con il virus per tutta la vita. Addirittura si arriva a una sieronegatività e quindi negli anni, fortunatamente, si è ridotto anche quello stigma sociale che avevano tutte le persone colpite dal virus HIV, perché è un virus che si riesce a tenere sotto controllo. Ma bisogna potenziare la prevenzione e bisogna lavorare molto di più sulla consapevolezza e sull'informazione, in particolare tra le giovani generazioni. Non è accettabile che

per un virus che invece, se diagnosticato in tempo, può essere tenuto sotto controllo. **Atti Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.